Il Presidente della Repubblica, con lettera del 9 settembre 2020, ha informato che, con decreto in pari data, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha nominato giudice della Corte costituzionale la professoressa Emanuela Navarretta. In data 12 settembre 2020 è stato presentato il seguente disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni

non rischi più fino a dieci anni e sei mesi di carcere, ma semplicemente - e solo forse - una sanzione amministrativa per essersi trattenuto i soldi della tassa di soggiorno, anziché versarli al Comune di Roma, di cui peraltro dovrebbe avere una certa fiducia essendo amministrato, come sappiamo, da un’esponente del MoVimento 5 Stelle. Mi sarei aspettato che ci fosse una richiesta del Presidente del Consiglio di venire a chiarire la situazione; invece, non solo non c’è richiesta, ma,

sollecito anche la risposta alle interrogazioni, a prima firma della senatrice Gallone, 4-03905 e 4-03999, sulla questione dei banchi di scuola:

per il singolo banco di 247,78 euro, quando su Internet io non sono riuscito a trovarne a un prezzo superiore ai 102 euro. Per comprarne uno!

spreco (che probabilmente un appartenente a un certo partito, molto battagliero sulle spese e sulla lotta agli sprechi, avrebbe chiamato ruberia) di 360 milioni di euro, come minimo, rapportando il costo al prezzo più alto reperibile su Internet. Trovo vergognoso che non vi sia risposta e trovo vergognosa la mancanza di trasparenza. Invito il Governo, che è qui autorevolmente rappresentato,

ha fatto un grosso favore al suocero con un provvedimento che dovrebbe essere di straordinaria necessità ed urgenza. Forse necessità e urgenza c’erano, ma la Costituzione si riferisce all’urgenza per lo Stato, non per i familiari, sia pure in famiglia informale. Atti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

con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (approvato dalla Camera dei deputati) - Relatrice